In data 10 dicembre 2010, il professor Ugo De Siervo ha inviato la seguente lettera: del 1953, che la Corte costituzionale, oggi riunita nella sua sede del Palazzo della Consulta, mi ha eletto Presidente. *F.to* Ugo De Siervo». Onorevoli colleghi, poiché è ancora in corso la Conferenza dei Capigruppo per la discussione del calendario dei lavori

A partire da oggi pomeriggio, alle ore 17, nelle due sedute di domani e, se necessario, venerdì mattina, sarà discusso il decreto-legge recante misure urgenti in materia di sicurezza, per il quale si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi. Gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 20 di questa sera.

2a devono convocarsi per proseguire i lavori alla presenza del Ministro. La prossima settimana, per l'esame del disegno di legge di riforma universitaria, l'Assemblea tornerà a riunirsi a partire da lunedì 20 dicembre in una seduta unica dalle ore 11 fino alle ore 21, con due sospensioni: alle ore 15, nonché, in relazione alla cerimonia di auguri al Capo dello Stato, dalle ore 16,30 alle ore 18,30. L'esame del disegno di legge sull'università si concluderà entro la seduta antimeridiana di mercoledì 22 dicembre e conseguentemente i tempi saranno ripartiti. Il calendario della prossima settimana

Presidente, come ho dichiarato a nome del mio Gruppo nella Conferenza dei Capigruppo, l'Italia dei Valori non è d'accordo con questo calendario. Apprezziamo un'ulteriore e approfondita discussione sul decreto-legge sicurezza e porremo anche al ministro Maroni alcuni interrogativi su quanto è successo nella giornata di ieri.

e che potrebbe aumentare nel corso di queste giornate, avevamo chiesto, e le chiediamo nuovamente in Aula, di avviare nella Commissione competente i lavori sulla riforma universitaria, ma di farlo in maniera cadenzata, dando rilevanza a tutte le istanze che ci sono e continuano ad esserci nel Paese, dagli studenti ai docenti, professori associati e anche agli stessi rettori, perché abbiamo bisogno che il Parlamento comprenda fino in fondo quali sono le difficoltà che questa riforma presenta e, se possibile, provando a correggere qualche errore che riteniamo contenga. Per queste ragioni, non ci vogliamo sottrarre ad alcun confronto, ma lo vogliamo fare

Presidente, come lei sa, noi non condividiamo il contenuto di questa riforma, ma questo, soprattutto in terza lettura, non è l'aspetto essenziale della nostra opposizione al calendario: lo dico per sgombrare il campo dal fatto che si possa pensare che la nostra contrarietà a questo calendario abbia in sé ragioni di natura meramente ostruzionistica.

La Commissione non ha ancora neanche cominciato ad esaminare un testo che reca 55 modifiche operate dalla Camera,

di spesa. Inoltre, come è noto, esiste nel Paese un movimento che conta centinaia di migliaia di ragazzi, di docenti, di ricercatori

Per questa ragione, ancora prima dei fatti accaduti ieri, ai quali - come è noto - gli studenti dissenzienti sono del tutto estranei,

dall'altra, se le modifiche apportate avessero incontrato o potessero incontrare il favore di quella grande parte del Paese che non condivide la riforma universitaria.

sul testo di riforma dell'università e che l'esame in Aula venga fissato per la prima settimana di ripresa dei lavori parlamentari dopo la sospensione per le festività natalizie.

dell'importanza di questo testo, delle modifiche che ad esso sono state apportate e anche di un movimento che si segnala nel Paese. Un attimo di riflessione e un tentativo di governo razionale, attraverso il confronto, avrebbero secondo me il potere di ricondurre il dibattito entro un ragionamento condiviso che valga ad assicurare al prosieguo dell'esame del disegno di legge di riforma dell'università un esito, affidato ovviamente alle maggioranze e alle opposizioni, e ai numeri che registreremo nelle Aule di Camera e Senato, e non invece ad uno scontro reso ancora più aspro da questa tensione sui termini di esame del testo.

del decreto-legge n. 187, in materia di sicurezza, su cui il mio Gruppo ha votato favorevolmente anche alla Camera, e soprattutto per quel pacchetto di norme antimafia che insieme ci siamo impegnati ad approvare,

Analogo ragionamento riguarda gli altri due provvedimenti concordati e inseriti all'ordine del giorno, per cui, dal nostro punto di vista, il calendario, per come è stato definito e ferme restando le nostre distinzioni e le nostre diversità di giudizio su alcuni provvedimenti, è accettabile.

di intervenire sul provvedimento. Dunque, credo sia giusta la calendarizzazione, fermo restando, ripeto, il confronto e il dibattito rispetto alle diverse posizioni che i Gruppi hanno espresso e manifestato sulla riforma. Queste sono le due motivazioni per le quali

anche noi condividiamo la proposta di calendario che lei ha formulato nella Conferenza dei Capigruppo e che adesso ha comunicato all'Aula.

per motivare la nostra adesione. Intanto valutiamo tutto l'insieme dei lavori che dobbiamo affrontare, a cominciare dall'intervento del ministro Maroni nelle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia che ci sarà tra poco, che agevola il percorso del decreto, che va convertito per la sua importanza, per la sua scadenza e per i suoi contenuti, e mi auguro agevoli anche un confronto politico-parlamentare su materie che da tempo sono all'attenzione del Senato, che sono state riassunte in ordini del giorno e che sono contenute anche nel disegno di legge che accompagna il decreto, e che ci siamo tutti impegnati a portare all'esame dell'Aula con la massima rapidità, nelle prossime settimane. Sulla vicenda sicurezza, mi pare che la discussione del decreto nei tempi previsti e la disponibilità del Governo e del ministro Maroni ad approfondire - e rispetto al decreto e rispetto

di atti internazionali - atti da noi condivisi e necessari, in taluni casi - dimostra che vi è stata una compilazione costruttiva e responsabile del calendario. Sulla riforma dell'università comprendo anche, dal punto di vista della dialettica politica, quanto detto da Gruppi di minoranza. Tuttavia, voglio ricordare che la riforma universitaria è stata lungamente discussa qui al Senato, dove

gli stanziamenti previsti, la tempistica che, a nostro avviso, suggerisce in maniera necessaria l'approvazione della riforma entro la fine dell'anno, la ricaduta del dibattito nel Paese, sia per i tanti che la riforma la auspicano,

un difficile ruolo nel Parlamento: se si decide, c'è tutta una serie di perplessità, se invece si allungano i tempi, veniamo considerati dei parlamentari che parlano senza discutere e senza decidere. Riteniamo che sia maturo il tempo per una terza lettura dell'Assemblea, che possa portare a delle decisioni, dopo mesi e mesi di ampio confronto nel Paese e nel Parlamento.

che fra l'altro è iscritto e militante del Partito radicale non violento, transnazionale e transpartito (ricordo che anche molti senatori in quest'Aula sono iscritti al Partito radicale), Partito radicale), è stato aggredito e picchiato dalla polizia della capitale della Mauritania, insieme ad un'altra trentina di militanti per i diritti umani, nel corso di una manifestazione che si teneva per la liberazione di due ragazze che sono ridotte in schiavitù presso un'alta esponente del potere locale (perché, forse non tutti sanno, ma in Mauritania ancora esiste la schiavitù).

di concerto con gli altri partner europei, avviare una decisa e forte campagna contro la schiavitù in Africa, a partire proprio dalla Mauritania. Oggi, sollecitiamo la risposta a questa interrogazione, insorta un'ulteriore preoccupazione, non avendo più notizie di Biram Dah Abeid: se ne sono letteralmente perse le tracce, e i nostri contatti in Mauritania

che non devono essere conosciute dagli elettori, posto che essi, purtroppo, non possono eleggere direttamente i loro rappresentanti in Parlamento. Tutto ciò servirebbe magari anche contenere nei limiti della decenza civile il rapporto tra i senatori; se ci fosse stata non soltanto la possibilità di pubblicità attraverso il canale radiofonico ma anche attraverso la televisione via Internet, che abbiamo, non così efficiente come quella della Camera, sul nostro sito «Senato.it», molto probabilmente avremmo potuto disporre di ulteriore documentazione su quanto accaduto ieri. Tra l'altro, ironia della sorte, una delle misure che avrebbe dovuto essere discussa ieri pomeriggio era la cosiddetta flagranza differita, che estende alle 48 ore successive la possibilità dell'arresto in flagranza, sulla base di documentazioni fotografiche e filmate. adottate con grande necessità e urgenza (se c'è un problema in Italia è quello delle manifestazioni sportive, dove sembra che succeda la guerra, mentre ieri mi sembra di aver capito che essa appartenga purtroppo ancora alle strade: ma se ne parlerà a mezzogiorno con il ministro Maroni), Maroni), occorre allora assumersi le proprie responsabilità e dare massima pubblicità ai nostri lavori. Ripeto, il Collegio dei senatori Questori ha espresso più volte parere favorevole in questa direzione. Non si capisce perché non si possa passare dalle parole ai fatti.

mi sembra totalmente insensata rispetto allo spirito di pubblicità che dovrebbe informare tutti i lavori parlamentari. Non si tratta di prevedere un obbligo di pubblicità, però di rimuovere quantomeno il divieto.

del ministro Maroni, ma vorrei sollecitare l'Aula a riflettere sul fatto che in due occasioni consecutive, in seguito a due votazioni fondamentali

della libertà italiana. Questi sono fatti gravissimi, che ci devono portare, al di là degli schieramenti, a riflettere, e anche ad agire. Quindi, era mia intenzione, e ne avevo parlato in maniera informale con altri colleghi, in particolare con i colleghi eletti nella città di Roma, presentare una mozione, la più ampia, la più condivisa e la più partecipata, che sottolinei la necessità che il Governo e le autorità competenti intervengano affinché sia scongiurato in futuro ogni tentativo di assalto al cuore della democrazia italiana. Io non ricordo episodi analoghi, neanche in Paesi del Sud America

cercare una condivisione, presentando una mozione con altri colleghi. In particolare, quest'anno festeggiamo i 150 anni dell'Unità d'Italia. Abbiamo promosso iniziative per Roma capitale, e io ritengo che Roma - il centro di Roma patrimonio mondiale dell'UNESCO - debba essere in qualche modo protetta da qualsiasi tipo di manifestazione.

è stato alimentato il conflitto sociale, e si è arrivati anche al terrorismo. Vorrei dire, signor Presidente, che non c'è alcuna giustificazione per degli studenti che hanno tirato

un Paese civile e democratico non possa accettare queste condizioni e che la reazione di un Parlamento che rappresenti la Nazione debba portare a condannare senza alcuna giustificazione questi gesti. Non erano studenti quei banditi che hanno attaccato le forze dell'ordine e hanno incendiato i mezzi di quei colleghi, di quei giovani che svolgono la loro professione professione difendendo le istituzioni dello Stato. Dico questo perché troppo spesso una certa cultura dell'omertà, o una certa cultura ideologica,

per far presente che ormai da molti anni (sia quando questo problema è stato posto dalle amministrazioni locali di centrosinistra, sia ora, in presenza di una Giunta di centrodestra) nella città di Roma è ben presente la preoccupazione di riordinare i meccanismi, le procedure, le condizioni attraverso i quali, democraticamente, si disciplinano le manifestazioni di dissenso o, comunque, in generale le manifestazioni politiche. il Ministro dell'interno, il Governo, la maggioranza - ma noi potremmo anche concorrere nelle sedi opportune - hanno ormai il dovere di immaginare che la Capitale non possa essere più soltanto il luogo dove ogni settimana, più volte alla settimana, si susseguono, arrecando un danno oggettivo alla sensazione di convivenza civile per tutti i cittadini di Roma, di Roma, grandi e piccoli eventi e manifestazioni di ogni tipo. Credo che la gestione dei grandi eventi e delle manifestazioni politiche dovrebbero fuoriuscire da questa condizione nella quale ciascuno, Comune e Stato, agisce con difficoltà in un contesto di coordinamento, ma ognuno con una precipua e limitata responsabilità. È giunto al momento di riordinare queste procedure e di fissare una cornice chiara. Anch'io considero inaccettabile qualsiasi tolleranza rispetto alla violenza che ieri si è perpetrata. Ho avuto modo di vedere chi erano coloro i quali partecipavano a queste manifestazioni con il volto coperto e con le spranghe in mano:

per manifestazioni che non colpiscono neanche un simbolo del potere *pro tempore*, cosa che già sarebbe inaccettabile, ma colpiscono le sedi della democrazia rappresentativa dove agisce sia la maggioranza

che si debba distinguere, come affermato anche dal senatore D'Ubaldo, tra chi si infiltra per provocare guerriglia, e che non deve avere cittadinanza (non basta la condanna: bisogna fare il possibile e l'impossibile perché questo non avvenga) e manifestazioni che sono espressione di legittima protesta, condivisa o meno, che si devono svolgere in modo pacifico e sul terreno civile. Bisogna pertanto tenere assolutamente divisi questi due aspetti. Nessuna incertezza e nessuna indulgenza nei confronti di coloro che usano la violenza

tutti noi dell'Italia dei Valori abbiamo espresso solidarietà e vicinanza alle forze dell'ordine. La ragione per la quale intervengo però è un'altra. Qualche giorno fa abbiamo appreso dai giornali nazionali ed internazionali che una cricca di banchieri gli amministratori delegati, i CEO, delle nove più importanti banche d'affari, da Goldman Sachs a Deutsche Bank - si riuniscono in segreto a Washington o a New York per decidere come indirizzare le speculazioni con i prodotti derivati, ossia come convogliare convogliare ingenti masse monetarie, create con la leva finanziaria, per colpire titoli del debito o obbligazioni degli Stati sovrani. Qualche giorno fa,

e le più prestigiose ed autorevoli banche d'affari del mondo invitavano gli operatori americani ed europei a disinvestire dalla Borsa italiana.

speculatori, di questi "bankster", che si arricchiscono per attentare alla sovranità degli Stati e alla ricchezza delle nazioni. Ricordo che, non noi, ma il direttore generale del Fondo monetario internazionale ha stimato in 30 milioni i posti di lavoro distrutti dalla speculazione dal 7 luglio 2007 (rammentiamo le file alla Northern Rock, eccetera).

e poi chi ci rimette è la povera gente, sono i lavoratori, gli impiegati, i pensionati, il potere d'acquisto. Non è possibile! Signor Presidente, io continuerò